Presidente, la scorsa settimana, abbiamo assistito ad uno spettacolo che non avremmo mai voluto vedere, e cioè al gesto inqualificabile del senatore Bettini. Siamo abituati nel dibattito parlamentare ad assistere a toni accesi, talvolta eccessivi, che però fanno parte della dialettica politica che sono proiezioni anche di quella passione che anima e muove la nostra azione quotidiana. Ma la volgarità, Presidente, non ha mai fatto ingresso nell'Aula di questo Senato e stupisce il silenzio della Presidenza, stupisce il silenzio delle parlamentari, delle senatrici della sinistra. Il gesto del senatore Bettini significa subordinazione intellettuale, significa subordinazione fisica e sessuale delle donne; è un gesto che lede la dignità personale, ancora prima della dignità politica: è un'offesa alle donne italiane. Qualcuno ha detto che questo gesto si giustifica come una reazione ad una situazione: io credo che la volgarità non sia mai una reazione; è un gesto che ha purtroppo una sua autonomia. Ed è per questo, Presidente, che è grave e deludente

contro la violenza domestica, per l'affermazione dei diritti delle donne. Anche questa è una forma di violenza ed è chiaro che chi combatte per la difesa dell'eguaglianza e della della democrazia ha posto come principio di riferimento la salvaguardia della dignità. Ed allora il silenzio delle parlamentari vanifica oggi questa battaglia comune, vanifica un comune lavoro

Chieda dunque il Presidente del Senato al senatore Bettini di rendere delle scuse formali a quest'Assemblea, chieda ai senatori e alle senatrici di chiedere scusa; diversamente, sembrerà a tutti - ce lo deve dire il Presidente del Senato - che in quest'Aula si possa fare qualsiasi cosa e che possa essere accolta perfino la vergogna. Prima di dare la parola ai senatori che me l'hanno chiesta, voglio ricordare ai colleghi che il presidente Caprili ha censurato non solo quello ora richiamato, ma anche altri episodi che si sono verificati che gli stessi sono stati riferiti al Presidente perché vengano discussi ed esaminati nella sede competente, che è quella del Consiglio di Presidenza. Io credo, rispetto a quella giornata, che frasi e gesti

dal Presidente di turno sia stata adatta e adeguata al clima per poter poi proseguire nei nostri lavori. Se qualcuno ora intende chiedere ancora la parola su quest'argomento, gliela

Gustavo Selva con lettera in data 11 giugno 2007. Il senatore Selva ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio anzitutto il presidente Altero Matteoli e l'onorevole Francesco Giro di Forza Italia, gli unici che si sono espressi pubblicamente sul mio caso dopo avere capito il significato politico delle mie dimissioni. In queste settimane, alcuni amici hanno giudicato che con le mie dimissioni io prendevo troppo sul serio l'"affare autoambulanza" (è vero che, nella storia di questa città, un'altra autoambulanza ha fatto - appunto - storia, 64 anni fa, in questo stesso mese; mi auguro almeno di non fare la fine dell'ospite di allora) o mi credevo io stesso troppo importante come bersaglio politico e massmediatico. Sarebbe così, onorevoli colleghi, se a scatenare la bufera non fossero stati tre aggettivi squalificanti con cui il ministro della salute, Livia Turco, senatrice, ha politicamente marchiato a fuoco il mio comportamento; i tre aggettivi squalificanti sono: "vergognoso", "irresponsabile", "indegno". Lasciamo stare i primi due, se vogliamo essere generosi; ma "indegno" vuol dire indegno di restare qui in mezzo a voi. Prese in assoluta solitudine, le mie dimissioni messe nelle sue mani, onorevole Presidente, erano la risposta che ho sentito il dovere di dare.

al Parlamento europeo, alla Camera dei deputati (dove ho assunto importanti ruoli istituzionali) e ora qui, al Senato della Repubblica, io ho fatto esclusivamente esercizio di parole scritte o radioteletrasmesse, cioè di idee; per cui davvero, con Carlo Levi, penso che anche stavolta le parole di una senatrice siano state pietre, che dovevano avere il loro seguito in quest'Aula, cosa che mi ci accingo a fare da parte mia. Anzitutto, i tre aggettivi hanno orientato i titoli e i commenti apparsi su tutti i quotidiani italiani e, nei giorni successivi, anche su gran parte della stampa e delle emittenti televisive internazionali. «*Le Monde*», con la penna di Robert Solé, ex corrispondente da Roma, ha scritto: «Perdere il posto per così poco è desolante. Se si pensa a tutte le ruberie, grandi o piccole, che permettono di accedere alle poltrone e di mantenerle, io mi rifiuto di gridare con il "commediante"». E, ironicamente, conclude con il detto italiano: «Non si spara sulla Croce rossa». C'era una soluzione immediata, onorevoli senatori, che avrebbe portato al ritiro altrettanto immediato delle dimissioni: era nelle mani del Ministro della salute per l'improvvida dichiarazione contro di me; l'avesse annullata quella dichiarazione, anche magari senza scusarsi, io avrei ritirato le dimissioni. Penso che la senatrice Turco non l'abbia fatto perché il Ministro della salute credeva forse di riequilibrare, con la sua accusa di indegnità, la bufera massmediatica che in quei giorni coinvolgeva - e per motivi ben diversi - i nomi di Fassino, D'Alema, Visco, i quali, giustamente, non hanno pensato neppure per un attimo a dimettersi, perché si trattava di materia su cui dovevano parlare per primi i giudici. Ma per loro nessuno, della destra o della sinistra, ha pronunciato la sentenza di indegnità di restare in Parlamento, come la senatrice Livia Turco ha fatto invece per me. Vediamo allora, se consentite, i fatti veri.

Invano. Il blocco era ferreo. Era tanto ferreo che anche un collega mi ha detto di non essere potuto entrare nella sua abitazione e questo sarà pronto a testimoniare. Le concitate telefonate mi hanno provocato fibrillazioni cardiache (non voglio la vostra indulgenza, ma sono portatore di quattro *bypass*), per cui sono stato accomodato e soccorso nell'ambulanza di servizio di Palazzo Chigi o di Palazzo Montecitorio. Sono stato poi trasportato all'ospedale San Giacomo. Mi sono ristabilito, forse anche in virtù del primo soccorso che mi sono dato io, che porto sempre il "Carvasin" con me, al punto che la Presidenza del Consiglio tenete presente, per favore, questo passaggio - mi proponeva una seconda macchina: è stata invece decisa, con il responsabile dell'autoambulanza, la soluzione di non mettere in moto un meccanismo ancora più complicato e di portarmi, con il mezzo in cui mi trovavo, in via Novaro. E qui, onorevoli senatori, si inserisce il fatto falso e disonorante per me, se fosse avvenuto, citato come principale motivo della mia indegnità dal ministro Turco: «Il bilancio poteva essere tragico nel caso in cui - e poteva accadere - un'altra persona avesse avuto realmente bisogno», realmente bisogno», parole della signora Turco (ANSA, 10 giugno 2007, ore 18,58). Questo "caso" non poteva, senatrice Turco, assolutamente accadere, perché quell'ambulanza era a disposizione esclusivamente di quanti, me compreso, che stavo assistendo alla conferenza stampa di Bush e Prodi, si trovavano nel cortile di Palazzo Chigi. Io c'ero, con regolare permesso. Le dichiarazioni del ministro Turco non sono state innocenti per me. Vi cito, fra le altre dello stesso tono, due *e-mail* ricevute lunedì 11:

schifoso maledetto!!!! Di cuore. Sei un imbecille, un arrogante, un ladrone della cosa pubblica per cui se vuoi salvare la Patria e il Senato (che purtroppo contiene altri a te pari) rinuncia alla tua carica e sparati un colpo in testa». Fin lì non ero disponibile in ogni caso ad arrivare. Le TV, le radio e i quotidiani, amplificando le dichiarazioni del ministro Turco, mi hanno "impiccato", per due giorni seguenti al fatto, quale "mostro di arroganza" del potere, con l'ingrediente, come ha scritto il quotidiano spagnolo «*El Mundo*» (che ho qui con me), di un "senatore della destra denunciato come indegno da un Ministro donna". Ne parlavano con toni critici quotidiani tedeschi e forse chissà di quali altri Paesi, con cui io ho avuto - ecco la mia sensibilità, se consentite - contatti ai più alti livelli politici e parlamentari, come Presidente della Commissione affari esteri della Camera dei deputati nella precedente legislatura, nella precedente legislatura, e con i quali continuo ad avere rapporti, quale componente della Commissione difesa, della Commissione politiche dell'Unione Europea e della delegazione parlamentare italiana Onorevoli senatori, le parole del ministro Livia Turco mi hanno addolorato, offeso, ma non meravigliato. Vedo che il lessico vetero-comunista, quando si tratta di usare la menzogna contro un avversario politico, è duro a morire anche in una senatrice *post*-comunista. Per conoscerci meglio con voi senatori della Repubblica, stiamo - se permettete per un momento - nel personale che, politicamente parlando - onorevole Presidente - è la mia storia giornalistica, culturale e civile: la storia della forte, reciproca battaglia democratica tra le mie idee di commentatore ed analista politico dei giornali e della radiotelevisione italiana e le idee comuniste, tradotte negli atti politici dei loro esponenti, da Togliatti a Longo, da Natta a Berlinguer, da decine di uomini di cultura, di giornalisti, di artisti e centinaia di migliaia di iscritti al Partito comunista italiano. Ero caporedattore per il Triveneto, negli anni '50, del quotidiano cattolico "L'Avvenire d'Italia" e ruppi, con un'inchiesta,

in Provincia di Treviso, dove furono prelevati dal collegio Brandolin 127 allievi ufficiali della Repubblica sociale italiana, di cui 80 massacrati dai partigiani comunisti, dopo che era stata firmata la resa il 28 aprile 1945, con la mediazione del parroco, monsignor Visentin. Quei giovani non avevano sparato un solo colpo né fatto alcuna operazione di guerra o di polizia; quei giovani richiamavano quello che io scrivevo ne "L'avvenire d'Italia", cioè quello che si chiama "gli orrori della guerra civile", di cui ci si ricorda oggi di più perché Giampaolo Pansa

Sempre sulla base delle menzogne o dell'alterazione dei fatti, fui il bersaglio di esponenti del Partito comunista italiano, de "l'Unità", di "Paese Sera", allora finanziato da Mosca, quando negli anni '60, corrispondente itinerante della RAI da Vienna per i Paesi del Centro e Sud Europa, appartenenti al blocco sovietico, ho documentato che i Partiti comunisti di quei Paesi controllavano con la polizia segreta ogni attività, ogni pensiero. Oggi questa è quasi un'osservazione banale di tutti i cittadini o quando ha trattato, ad esempio, nel mio lungo documentario televisivo, la donna che lavora nell'Est, dell'impiego delle donne nelle fabbriche, nelle campagne, nella polizia notturna delle strade a 30 gradi sotto zero. L'Unità ha scritto, sulla base della dichiarazione dell'onorevole Pajetta, che offendevo le conquiste del socialismo e della parità tra uomo e donna. Durante la prima *Grosse Koalition* in Germania, dopo il '68, analizzavo analizzavo l'APO - *Ausserparlamentarische Opposition* - extraparlamentare di Francoforte e di Berlino Ovest - so che sapete a memoria tutto questo; le richiamo me stesso, come dicono gli avvocati; quindi non avete bisogno di ascoltarmi con attenzione. Le conoscete tutte così bene tanto perché le avete spiegate così bene quando a quei tempi queste avvenivano! - come centri operativi delle violente manifestazioni contro Willy Brandt ed ancora più contro Franz Joseph Strauss, presentato come neonazista. L'APO fu da me indicata ai teleradioascoltatori italiani, nelle mie corrispondenze per la radio e la televisione, come il brodo di coltura da cui sarebbe nato la Rote Armee Fraktion e per tutto questo "l'Unità" mi dipingeva come un fautore della guerra fredda e un sostenitore dell'imperialismo americano. La storia del Gr2 - ho piacere che sia qui presente come mio collega il senatore Sergio Zavoli, che ne potrà dare testimonianza - è troppo nota per essere però ricordata soltanto come "Radio Belva",

necessario). In quei commenti e soprattutto nei miei editoriali mi sembra di aver indicato le vie attraverso le quali gli stessi comunisti del Partito comunista italiano avrebbero dovuto e potuto, prima della Bolognina dell'onorevole Occhetto, rinunciare ai miti

applicato o di quello che voi chiamavate il socialismo reale, cioè, impegnarvi, come poi il Partito comunista ha fatto, alla costruzione dell'Unione Europea, più giusta e solidale, della collaborazione euroatlantica per la garanzia di pace e di libertà.

nell'elenco della P2 (documentata oltre che da tre commissioni anche dalla mia vittoria in un processo per diffamazione contro Dario Fo, e che è stata presentata in un comunicato quando io sono stato estrapolato dalla direzione del Gr2

e l'accordo consociativo fra i consiglieri di amministrazione comunista e della sinistra democristiana della RAI, che determinarono la mia defenestrazione dalla direzione del Gr2. fondata, ripeto, sull'apodittica definizione "comunque coinvolto", che, ripeto, non so francamente ‑ non sono avvocato ‑ che cosa voglia dire. La mia risposta fu molto chiara e anche in questo Sergio Zavoli, che allora presiedeva la RAI, me ne è testimone. Io risposi al microfono per spiegare ai miei ascoltatori, che erano andati sempre più aumentando, quali erano le ragioni per cui mi avevano defenestrato. La ragione vera è quella, onorevoli colleghi, di essere stato, specialmente nei miei editoriali, l'autore di una linea politica che in RAI non c'era e che scoprì prima di Rossana Rossanda che nell'album di famiglia del PCI e nelle manifestazioni katanghesi di Milano contro il commissario Calabresi c'erano intellettuali del PCI e quadri operativi della sinistra, che oggi si chiamerebbero forse antagonisti, alcuni dei quali, negli anni Settanta fecero la scelta del Partito comunista combattente, delle Brigate Rosse o di Prima Linea, con la catena di assassini di servitori dello Stato, dai Carabinieri ai poliziotti,

a dirigenti politici, in prevalenza democristiani, fino all'attacco al cuore dello Stato portato dalle Brigate Rosse con l'assassinio di Aldo Moro.

Onorevoli senatori, colgo in positivo, in una vicenda che mi amareggia, il campanello di allarme che suona per tutti noi come per me, mai toccato da fatti giudiziari che riguardassero corruzione, concussione, furto, tangenti, malversazioni, aggiotaggio, bancarotta, associazione mafiosa, spaccio e consumo di cocaina. Mai nessuna di queste responsabilità penali mi ha toccato. Non commettiamo l'errore, onorevoli senatori, di liberarci dalle critiche, anche se pregiudiziali, che ci coinvolgono, dando loro la definizione assolutoria di anti politica. Il rispetto del valore insostituibile della democrazia liberale al servizio del cittadino sarà riconosciuto se anche gli uomini e le donne della politica, cioè noi, qui ed ora nelle istituzioni italiane affrontiamo realmente anche i costi e i privilegi che la politica si è assegnata. Dobbiamo fare delle istituzioni, onorevoli senatori, e specialmente di quelle elettive, una casa di vetro, non opaco però, nella quale operi non una casta, bensì donne e uomini, e in maggioranza sono questi, dediti alla promozione e alla difesa dei valori etici, civili, religiosi, umani di ogni cittadino. L'uscita dal Senato, onorevoli senatori, sarebbe per me la bella morte politica di un eroe per un giorno dopo l'ondata dei messaggi insultanti del tipo di quello letto all'inizio. Cessata l'esposizione mediatica del mio nome, su cui tutta la stampa ha fatto silenzio, anche quando io ripetutamente chiedevo, per dire queste cose, che venisse messo all'ordine del giorno quanto è oggi all' ordine del giorno del Senato, da parte di ogni città di Italia, soprattutto dal Veneto, mio collegio elettorale, sono arrivati tantissimi messaggi che mi invitano a restare. Nel Veneto, io ho conquistato per Alleanza Nazionale un seggio che non c'era. Sono, quindi, un numero in più per la Casa delle libertà che ha ritrovato, anche per le mie idee per il mio impegno politico culturale, nel primo caso come giornalista e nel secondo come parlamentare, uno che avvicina il numero dei senatori dei Gruppi dell'opposizione della Casa delle Libertà a quella quota della maggioranza dell'Assemblea della maggioranza di Palazzo Madama. Prima o poi, Romano Prodi cadrà, per opera dell'opposizione o, forse, a causa dei durissimi programmatici esistenti fra i ministri. Nel partito democratico stesso, fra i vari candidati, sarà una bella battaglia per fare di Veltroni un candidato imbattibile visto che già due altri concorrenti, Rosy Bindi e Furio Colombo, al quale formulo i migliori auguri, sono scesi in campo per mettere in rilievo, credo, anche le contraddizioni del programma torinese. L'unica cosa certa del partito democratico, e lo dico a me stesso, è la scomparsa di ogni identità cattolica. Onorevoli senatori, il pensiero che un voto in meno del centro‑destra possa concedere un giorno in più al Governo Prodi travolge ogni altra ragione che mi spingerebbe alle dimissioni. Mi spiace per il ministro Livia Turco, ma più delle sue accuse mi interessa il giudizio sereno di tanti cittadini che in questo lungo mese mi telefonato e che ho incontrato, specialmente nel Veneto così come nelle strade. E sono tutti messaggi che mi invitano a restare. Assumo su di me la responsabilità politica di ritirare le dimissioni presentate con lettera dell'11 giugno.

di agenzia che dice: «Il neoprocuratore aggiunto Pierfilippo Laviani ha concluso l'inchiesta che vede indagato per accuse di truffa

perché se un'assoluzione dovesse venire da voi potrebbe sembrare la casta che si autodifende. Non voglio darvi questa responsabilità.

con un bipolarismo che non sia né solo «follinianamente» mite, né formato da pure coalizioni per vincere le elezioni.

L'alternanza garantita da programmi politici omogenei è il sale della democrazia, prima che le caste di partito sarà bene che nel *referendum* ascoltiamo che cosa pensano i cittadini della legge elettorale. In Europa, in Francia si è costruito un bipolarismo che funziona. Forse anche per noi è necessario che ci siano, insieme con la nuova legge, delle riforme istituzionali che rendano la quinta Repubblica anche governabile e modernizzata. Senatore Selva, non voglio toglierle la parola; quindi, non mi costringa a farlo. SELVA *(AN)*. Io mi batterò qui per i valori della sicurezza interna e internazionale dei popoli che aspirano alla libertà, alla giustizia, alla pace, la difesa di quei valori etici di ogni persona e della famiglia, come definita dall'articolo 29 della nostra Costituzione, che io proporrò di perfezionare aggiungendo dopo la parola «matrimonio», le parole

Signor Presidente, in meno di un minuto vorrei poter aiutare questo Senato a meglio comprendere le ragioni

che, dai tempi di Cicerone e delle sue «Filippiche», è abituato a toni aspri, non sempre mediati da eleganza di linguaggio, ma non per questo meno importanti. Forma e sostanza qualche volta si confondono ed io chiedo scusa a quest'Aula soprattutto per non aver contribuito a quel chiarimento e a quel giudizio sereno che innanzi tutto qui, qui, come nell'altro ramo del Parlamento, dovrebbero accompagnare il dibattito sulla giustizia che invece resta, ahimè, sempre vittima di posizioni precostituite e di tante ferite che il Paese porta ancora con sé, tutte aperte.

per me sono il controcanto e il contraltare di una giustizia nella quale non dobbiamo mai perdere la fiducia e verso la quale dobbiamo avere atteggiamento attento e sereno di collaborazione. il procuratore Guido Papalia, secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera» di domenica, ha detto: conosco bene la senatrice Bonfrisco, so quanta correttezza ed equilibrio guidano il suo lavoro; deve essere successo qualcosa in quell'Aula che ha riaperto antiche ferite e deve averla provocata. Quello che è successo a me è successo a tanti altri cittadini. Da domani, quando con serenità si potrà riprendere questo dibattito, nello specifico sulla storia

Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Non ho avuto modo, purtroppo, di ascoltare all'inizio della seduta se è stata data notizia, da parte della Presidenza dell'Assemblea, dei lavori della Conferenza dei Capigruppo. Ho motivo, però, di ritenere che la cosa di cui desidero informare i colleghi, con tutta la riservatezza necessaria, riguardi la questione molto delicata posta dai colleghi Manzione e Bordon

Signor Presidente, avevo chiesto la parola, perché pensavo che oggi si discutesse delle dismissioni del senatore Gustavo Selva

circa 40 minuti, nel quale il suddetto senatore Selva ha fatto la propria autobiografia, nonché una requisitoria contro la sinistra nella storia italiana, nonché un attacco continuato ad una Ministra del Governo in carica, apprendo, con un *coup de théâtre* finale (del resto molto annunciato e previsto), che il suddetto senatore ritira le proprie dimissioni. Naturalmente, non discuto il suo diritto, né l'opportunità che il gesto offre ai colleghi del centro-destra di mantenere la certezza di un'unità del proprio schieramento,

di un episodio inqualificabile di uso per scopi privati e frivoli e personali di un'autoambulanza, di dichiarazioni farneticanti sui giornali e di rivendicazione esplicita

che quest'Assemblea dovrebbe avere a cuore più di ogni altra cosa: egli offende la dignità e la serietà della politica e delle proprie responsabilità. Presidente, viviamo in un'epoca in cui tutta la politica vive una fase difficile. C'è una dura campagna critica contro l'intera classe politica, contro i privilegi, i costi e, appunto, la bruttezza di ciò che noi rappresentiamo. Credo che sia un problema molto serio per tutti noi. Ritengo che non riguardi, quindi, semplicemente i singoli: riguarda tutti i comportamenti dei dei singoli colleghi, di qualunque schieramento facciano parte; riguarda tutti noi perché c'è un punto fondamentale di dignità, di serietà e di responsabilità che riguarda la qualità della politica e la responsabilità che noi

si toglieva qualsiasi limite alle grandi imprese che si occupano di distribuzione e vendita di energia per fornire servizi anche nel cosiddetto post-contatore. Con la legge Marzano nella passata legislatura si misero paletti ben fermi - Alleanza Nazionale fece una battaglia in questo senso - proprio a tutela delle imprese artigiane per favorire la concorrenza, che sarebbe impedita da situazioni di monopolio che in tutta evidenza che in tutta evidenza danneggiano, in primo luogo, l'interesse del consumatore. Ora, con la legge Bonino il Governo ha ripristinato la discriminazione di sette anni fa. In realtà, occorre capire se si vogliono privilegiare i grandi interessi - soliti referenti del centro‑sinistra, i grandi gruppi oligopolistici; oligopolistici; penso alla storia che si ripete, al caso Telecom, che in qualche modo si ripete - anziché difendere la rete diffusa della nostra produzione artigianale. Credo che la sinistra debba dare una risposta su un tema così delicato ed importante. Tutte le Confederazioni - dalla CNA, alla Confartigianato, all'Unione artigiani - si sono espresse nella direzione rappresentata da questo emendamento.

ad evitare situazioni di sostanziale monopolio e a provvedere nel senso recepito da questo emendamento. Quell'ordine del giorno venne accolto dal Governo, che si impegnò a modificare il testo della legge Bonino. Vorrei dunque capire ora abbiamo la possibilità concreta di comprendere - se il Governo considera gli ordini del giorno pezzi di carta straccia, senza alcun valore e senza alcuna conseguenza,

per assicurare l'obiettivo dell'accesso ai dati trovino copertura attraverso la previsione da parte dell'Autorità

si vuole consentire a più produttori di condividere, oltre alla rete di distribuzione, anche la rete di adduzione. Attualmente, se due produttori, per esempio di energia idroelettrica, sono contigui, debbono realizzare due linee di adduzione

Presidente, a seguito del voto favorevole sull'emendamento del relatore 1.206, una serie di emendamenti da me presentati come primo firmatario sarebbero stati considerati assorbiti, ma

Signor Presidente, pur riconoscendo senz'altro la necessità e l'urgenza del provvedimento per quanto riguarda il settore elettrico, a nostro avviso non si ravvisa la stessa necessità per il settore del gas, che deve essere trattato ben diversamente e con maggiore attenzione.

carenza di recepimento nell'ordinamento legislativo delle disposizioni di cui alla direttiva europea n. 54 del 2003.

vigenti anche in Italia. Tale adozione di uno o più decreti legislativi, prevista a partire dal 18 aprile 2005 per la durata di un anno, non si è verificata per un motivo o per un altro. Nessuno dei Governi che si sono succeduti da allora ha ritenuto di adottare i decreti legislativi. In conclusione, siamo in carenza di applicazione di varie disposizioni di questa di questa direttiva comunitaria. La motivazione del decreto‑legge è proprio quella di far fronte, essendoci una serie di osservazioni nell'ambito di una procedura di infrazione

Tale direttiva riguarda unicamente l'energia elettrica; allora, perché inserire in un decreto-legge, che effettivamente è adottato per venire incontro ad esigenze di straordinaria necessità ed urgenza

1 dell'articolo 1, che prescrive la separazione funzionale delle imprese che effettuano lo stoccaggio di gas. La separazione societaria vi è già perché vi è un'unica società in Italia che cura lo stoccaggio del gas, la Stogit SpA del gruppo ENI. La separazione funzionale penso ci sia già di fatto; quindi, non ci sono elementi di contrasto rispetto a questa disposizione nel contenuto.

clienti sono di proprietà dei clienti stessi, e fin qui ci siamo. L'emendamento che ho proposto subordina l'accesso di terzi a questi dati all'acquisizione esplicita del consenso di coloro che sono titolari dei dati le norme in materia di *privacy* stabiliscono che è unicamente il titolare dei dati personali ad avere la competenza e a decidere sulle finalità, le modalità e l'impiego

dopo le parole «comprendono tra le proprie offerte commerciali», inserire le altre «contemplando anche la possibilità di scegliere tra piani tariffari e fasce orarie differenziate

essere risarcite economicamente, ma richiedono una particolare attivazione di strumenti energetici; pensiamo a tutti coloro che sono legati a macchine o a particolari condizioni di asma bronchiale. Vorrei chiedere al relatore se si tratta di una svista o se magari, nelle condizioni

Presidente, sono costretto a ripetermi nel pregare il relatore e il Governo a darmi una risposta sul termine «transitoriamente», al rigo terzo dell'emendamento

di tipo inquisitorio, così io chiedo in questo momento all'Aula, in particolare al relatore e al rappresentante del Governo, come si fa in tredici giorni a cambiare completamente opinione e qual è la coerenza coerenza nell'usare il termine «transitoriamente», che in Italia vuol dire "definitivo", perché tutte le cose che si fanno transitoriamente non si modificano più. Non mi sembra serio che un provvedimento che è stato discusso approfonditamente in Commissione venga poi stravolto per ordini esterni, visto che al riguardo io stesso ho ricevuto proteste di carattere sindacale. Allora, ritengo debbano essere seri il relatore e il Governo nel dare una risposta.

affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di determinare condizioni *standard* di erogazione dell'energia elettrica. È una

che non ha i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Non si vede per quale motivo debbano essere definiti questi prezzi di riferimento. In secondo luogo, non si comprende come l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in una situazione di totale affidamento al mercato, dal 1° luglio 2007, possa stabilire questi prezzi di riferimento, sia pure per i clienti finali domestici. Come fa a stabilirlo? Tra l'altro, nel testo è scritto: «in base ai costi effettivi». Ma quale *markup* sui costi effettivi può permettersi di inserire l'Autorità per l'energia elettrica e il gas? Con quali criteri? Credo che ciò sia totalmente impossibile. Inoltre, il prezzo dell'energia elettrica, per effetto della struttura di mercato che vale ormai per tutti i clienti dal 1° luglio 2007, è determinato dal mercato stesso ora oltre che giorno per giorno. Non è prevedibile *ex* *ante*. Come fa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad affrontare ciò, sia pure transitoriamente?

un termine di ragionevole cautela per una fase transitoria. Comunque mi sembra che, pur con la dolcezza dell'avverbio «transitoriamente», il Governo esprima in questa circostanza una certa diffidenza sul funzionamento di mercato. Vi è un ultimo aspetto che vorrei segnalare all'attenzione sua, signor Presidente, e dei colleghi, in particolare a quella del Presidente della Commissione bilancio.

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di svantaggio economico». Mi chiedo, signor Presidente, chi paga e se è previsto - mi rivolgo al Presidente della Commissione bilancio

la remissione alla Commissione da parte del Governo. Questi emendamenti - approvati dall'intera Commissione all'unanimità - eliminavano l'obbligo di inserire il prezzo di riferimento nelle offerte commerciali e rispondevano meglio, quindi, all'effettiva liberalizzazione del mercato.

proprio per gli aspetti fondamentali per cui il lavoro effettuato in Commissione non va vanificato in Aula, saremo costretti a votare decisamente contro questo provvedimento.

Vorrei semplicemente svolgere due considerazioni rispetto agli argomenti usati dal collega Possa e dal collega Maninetti. Questo è stato il punto più discusso durante il dibattito in Commissione: sul merito del decreto la Commissione ha avuto, nella sua unanimità, un atteggiamento positivo, ma la questione dei prezzi di riferimento è stata quella sulla quale si è sviluppata la discussione più approfondita. Non vi è mai stata una differenza di impostazione su questo perché anche chi ha approvato l'emendamento in discussione, adesso riformulato in questo testo, è dell'idea che i prezzi di riferimento siano un elemento un elemento transitorio e dedicato ad una porzione limitata dell'universo dei cosiddetti clienti, oggetto del provvedimento. Da questo punto di vista, è ricondotta ad una dimensione molto più limitata anche la portata degli argomenti argomenti di opposizione, qui richiamati. Il termine "transitoriamente" è stato utilizzato proprio per mettere in evidenza questo concetto: stiamo parlando di un istituto, il prezzo di riferimento, che ha un valore temporaneo che, ovviamente, può anche essere inferiore ai due anni proposti in alcuni emendamenti, ma che serve ad accompagnare con equilibrio il processo di liberalizzazione, così come viene proposto. Un'ultima osservazione, con riferimento alle fasce

attuato una piena liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. I clienti domestici e le piccole imprese assimilate ai clienti domestici possono, di fronte a questa piena liberalizzazione, avere delle difficoltà. È opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettui per un periodo limitato di tempo, appunto due anni, una vigilanza su questo passaggio, dopo di che sarà il mercato a decidere i prezzi dell'energia elettrica; il mercato, sapendo bene di avere costruito una struttura competitiva, contendibile, garantirà

prima che lei mi dica, che il successivo emendamento 1.208 è stato eliminato per altre ragioni, mi permetto di farle notare che esso è un corpo estraneo, un autentico clandestino a bordo, in quanto non si riferisce al disegno di legge n. 1649, non so francamente come sia stato accettato dagli Uffici, ma al disegno di legge n. 1644 sulle liberalizzazioni.

molto esaustiva anche all'interno della Commissione. È vero che si è raggiunto un accordo, ma credo che l'avverbio «transitoriamente» dia l'idea di come si creda o no alla liberalizzazione. Credo che deve essere il mercato a deciderlo e condivido, come ha detto il collega Cabras, che i due anni possono essere un limite che va oltre le esigenze del mercato.

cercano di portare verso una vera liberalizzazione, salvaguardando, comunque, realmente, i clienti domestici, ponendo un chiaro limite ai consumi. Gli emendamenti escludono

cospicua sfiducia nei riguardi del mercato. Lo leggo per chiarezza mia e dei colleghi: «Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. Questa sottolineatura dei poteri che comunque ha, per la sua legge istitutiva, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta in questi termini,

Per tale motivo, propongo la soppressione di quelle righe, totalmente pleonastiche perché l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha già il suo mandato stabilito

chi dobbiamo ascoltare e chi comanda, perché ho l'impressione che noi si comandi un po' poco. Deliberiamo sulla giustizia e dobbiamo ascoltare molto attentamente l'Associazione nazionale magistrati,

signor Sottosegretario, è quando i prezzi in Russia li decideva il *Politburo*, per cui c'era tutto allo stesso prezzo nella stessa parte. Ma allora perché dobbiamo mantenere la borsa per l'energia elettrica, perché dobbiamo mantenere le contrattazioni, perché dobbiamo mantenere l'acquirente unico, che in qualche modo svolge un'operazione di *benchmarketing* e fissa anche un *price cap*?

Già oggi il prezzo dell'energia elettrica e del gas deve rispondere ad una serie di misure, per cui c'è una componente dei costi della trasmissione e della distribuzione:

della fascia media dei consumatori, quindi della piccola e della media impresa. Ricordo che un'impresa media italiana paga di energia circa venti volte in più del corrispettivo tedesco, quindi, quando parliamo di competizione e quant'altro, dobbiamo ricordarci che le imprese energivore delle altre parti d'Europa sono estremamente competitive. Se per la prima fascia abbassiamo i costi, che può anche essere condivisibile, dobbiamo anche precisare per chi li andiamo ad aumentare. Per questi motivi, dichiaro il voto contraria della Lega Nord

Questo è un Parlamento menomato, perché in realtà riceve ordini dall'esterno. Quattordici giorni fa alcuni colleghi hanno votato in un modo, adesso subiscono questo *diktat* del relatore e del rappresentante del Governo. Questo è un Parlamento che ha le mani legate,

giorni per adempiere a tutte le disposizioni previste dal decreto-legge sono assolutamente non sufficienti. In effetti, in Commissione avevamo deciso novanta giorni.

sia il Governo sia il relatore non vogliano accettare l'emendamento 1.0.100, che è nello spirito della liberalizzazione. Insomma, si tratta di condividere una linea elettrica; capisco la posizione dell'ex monopolista, ma siccome stiamo parlando di un sistema libero, il monopolista non c'è più e non vedo perché non si debba condividere la rete di adduzione. Chiedo

Ove la discussione del decreto-legge in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia - per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi - dovesse concludersi prima delle ore 20,30, l'ordine del giorno sarà integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge comunitaria, che proseguirà nella giornata di domani. Su richiesta del Governo, il seguito del disegno di legge in materia fiscale è rinviato a una data successiva all'esame del decreto-legge in materia finanziaria - attualmente in discussione alla Camera dei deputati - che ne anticipa alcune misure. Sempre su richiesta del Governo, l'esame del disegno di legge n. 691, recante delega per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas - di cui il decreto-legge all'ordine del giorno di oggi anticipa alcune norme - avrà luogo a settembre, alla ripresa dei lavori. Il calendario della settimana comprende poi la discussione generale del disegno di legge di riforma del sistema di informazione e sicurezza, ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, compresa la ratifica con l'UNESCO, e il disegno di legge sulla ricostituzione di fondi e banche internazionali. Gli emendamenti al richiamato disegno di legge di riforma del sistema di informazione e sicurezza dovranno essere presentati entro le ore 19 di domani. Le votazioni potranno iniziare a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 24 luglio. Per quanto riguarda il dibattito di politica estera, sollecitato da alcuni Gruppi con particolare riferimento alle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri ha manifestato il proprio orientamento a rendere comunicazioni al Senato nella seduta pomeridiana di martedì 24. Di ciò sarà data tempestiva conferma ai Presidenti dei Gruppi. La successiva discussione potrà concludersi con votazione di strumenti di indirizzo. Mercoledì 25 luglio sarà discusso il Documento di programmazione economico-finanziaria. La prossima Conferenza dei Capigruppo procederà alla ripartizione dei tempi ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Seguirà l'esame del disegno di legge delega per il riordino dei servizi pubblici locali. Infine, i Capigruppo hanno manifestato la propria disponibilità al trasferimento in sede deliberante per le norme del disegno di legge n. 1598 in materia di professione intramuraria, in corso di esame presso la 12a Commissione permanente. Per quanto riguarda la lettera inviata dai senatori Bordon e Manzione con riferimento all'articolo 67 della Costituzione, la Presidenza si è riservata di procedere a un opportuno approfondimento.

sulla conferenza stampa del ministro Bonino, la quale - sempre secondo alcune agenzie - avrebbe rimesso il mandato nelle mani del presidente del Consiglio Prodi.

né è la prima volta che un Ministro si dimette perché non condivide un provvedimento. Anche in questi giorni abbiamo assistito in quest'Aula agli interventi

valuti lui - il Presidente del Consiglio ‑ se è compatibile il nostro sostegno al Governo, visto che siamo una formazione riformatrice, determinata su questi temi.

tra un'area massimalista e un'area riformista. È dunque uno scontro politico di grande rilevanza, stando alle motivazioni del ministro Bonino. Chiedo quindi al Governo se non intende venire a riferire immediatamente su questo argomento per capire se il presidente Prodi ha intenzione di prendere una posizione a favore della politica riformista o di quella massimalista,

del senatore Matteoli, il quale, molto correttamente, ha ricordato che si tratta di agenzie di stampa che indicano una volontà da parte di un Ministro della Repubblica. Quindi, io credo che questa sollecitazione sia assolutamente giusta e e la riferirò al presidente Marini perché valuti la possibilità di acquisire tutte le notizie del caso, che ancora sono sotto forma di comunicati stampa,

ed in particolare a quella parte delle comunicazioni che riguardano una prima risposta alla lettera che ieri io e il senatore Manzione abbiamo inviato al presidente Marini. Ovviamente, non avendo ancora se non una risposta di carattere interlocutorio, se ho capito bene, per approfondire più accuratamente i problemi che quella lettera poneva, non posso intervenire nel merito di una questione non ancora risolta, almeno per quanto riguarda la Presidenza. Voglio soltanto specificare, perché vorrei che non ci fossero dubbi che la questione non riguarda, come è evidente - altrimenti, francamente, non meriterebbe l'attenzione né il tempo perso da parte di questa autorevole Assemblea - il cosiddetto caso Bordon‑Manzione che, fra l'altro, come si è visto,

ce ne potrebbero essere, ce ne saranno e ce ne saranno anche state probabilmente altre - del dibattito parlamentare, metteva in luce il rapporto sempre più delicato che c'è fra l'articolo 67 della nostra Carta costituzionale, che, come sapete, non pone limiti allo svolgimento della propria attività parlamentare, al proprio mandato, se non l'interesse esclusivo della Nazione (come recita testualmente), e il Regolamento ed eventualmente le misure disciplinari dei Gruppi parlamentari stessi. Tale questione, sia ben chiaro, è delicatissima - ne parlavo prima con il senatore D'Onofrio - e presenta tratti non facilmente definibili*tout court*, ma a mio avviso ha una caratteristica oggi invero assai particolare. Infatti, noi non possiamo ignorare che c'è una differenza oggi nella determinazione delle platee parlamentari, che con la nuova legge elettorale sono, come sappiamo, sempre di più per molti versi designate, se non nominate, dalle segreterie dei partiti. Quindi, è evidente come si possa creare un corto circuito non facilmente risolvibile, nel momento in cui, con questa legge elettorale, il singolo parlamentare può trovarsi in una condizione di preoccupazione, lecita e comprensibile, rispetto ad una sua eventuale ricandidatura in una lista bloccata, rispetto al suo diritto e alla sua prerogativa fondamentale (vorrei ricordarlo), perno di una democrazia liberale e della nostra Costituzione. Il problema pertanto non può essere affrontato, a mio avviso, soltanto nel ristretto dibattito di questo o di quel Gruppo parlamentare, ma merita di essere affrontato in quest'Aula. Insisto quindi perché lo si faccia spero che la Conferenza dei Capigruppo vorrà accettarlo anche perché, memore anche di alcuni interventi che feci quando svolgevo il ruolo di Capogruppo di opposizione, vorrei ricordare che questioni del genere non attengono all'interesse di questa o di quella parte ma dovrebbero essere affrontate con quello che un grande pensatore e filosofo liberale americano definiva

ci dovessimo rendere conto che in effetti la libertà prevista dall'articolo 67 viene di fatto messa in discussione da interpretazioni troppo rigide della disciplina dei Gruppi parlamentari, sia bene parlarne in

quello di oggi è un primo, importante passo per un diverso modello energetico, capace di coniugare sviluppo, diritti degli utenti e dei cittadini e ambiente. Noi sosterremo con convinzione questo provvedimento, non solo perché rafforza il potere di acquisto delle famiglie e riduce intollerabili rendite, ma perché, se correttamente orientato, è una grande opportunità per la sostenibilità ambientale e per raggiungere quegli inderogabili obiettivi, fissati pochi mesi fa dall'Unione Europea, di una riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2020. Quello che compiamo oggi è un primo passo verso un modello di vasta portata, coerenti con gli impegni che l'Unione Europea ha preso. Auspichiamo pertanto che questo disegno normativo complessivo possa presto pienamente definirsi. Spero sia consapevolezza diffusa in quest'Aula che i tasselli ancora mancanti non devono venire meno né dall'agenda del Governo né dall'agenda del Parlamento. Non possiamo infatti non rilevare come proprio al Senato giaccia, ormai all'ordine del giorno dell'Aula da settimane, una proposta di delega più complessiva, che avrebbe consentito, ove approvata in maniera più celere, di far collimare questi due tasselli: da un lato, un mercato libero e aperto, dove i cittadini possano godere, alle migliori condizioni e responsabilmente, di fonti energetiche sicure; dall'altro, un cambiamento profondo dei modi di produrre energia. Questi sono i due pilastri su cui poggia questo disegno normativo complessivo: mercato e sostenibilità ambientale, quindi economia ed ecologia.

e che imporre regole di concorrenza in comparti dominati dai monopolisti significa consegnarsi alle rendite. Questo è stato il punto di frizione sui prezzi di riferimento in Commissione. Ritenere che basti una legge a dare vita ad un mercato libero è, purtroppo, un atteggiamento inadeguato, che non tiene conto del fatto che la denazionalizzazione è un processo complesso che dev'essere orientato nella direzione dell'interesse generale. Servono regole graduali, che consentano la rivoluzione culturale nella produzione di energia e la liberalizzazione nella distribuzione. E questo deve avvenire dentro il sistema Europa: la sfida energetica non può essere vinta da un solo Paese. EUROSTAT ci dice che oggi, in Europa, il 60 per cento dell'elettricità è prodotta da fonti fossili, il 20 per cento dal nucleare e che, se escludiamo la fonte idroelettrica, ormai satura, le fonti rinnovabili incidono solo per meno del 5 Con lo sblocco delle risorse destinate alla ricerca connesse agli oneri generali, possiamo dare forza anche all'altro pilastro: riavviare l'impegno pubblico in ricerca, soprattutto per le energie rinnovabili, che ci consentirà di colmare un ritardo profondo. Questo Paese ha sperperato 13 miliardi di euro in dieci anni per sostenere fonti fossili ed inquinanti, sottratti con un prelievo forzoso dalla bolletta dei cittadini, attraverso l'alibi che quelle risorse fossero destinate a fonti rinnovabili, contro la normativa europea. È uno scandalo noto, ormai alla luce del sole. Nonostante questo, tanti nomi italiani importanti a livello internazionale sono cresciuti nel campo delle energie fotovoltaiche, del solare termodinamico, delle biomasse di origine agricola. E nuove stimolanti prospettive abbiamo da territori di frontiera, come è la geotermia profonda. Sono questi gli elementi di un disegno di cui questo provvedimento è un tassello estremamente rilevante. A chi pensa alla liberalizzazione in campo elettrico solo come alla competizione tra grandi campioni nazionali che si sfidano sul nostro territorio, magari senza troppo rispetto per i luoghi dove operano, noi oggi suggeriamo un modello diverso, quello che migliaia di famiglie stanno in questi mesi sperimentando con il conto energia sul fotovoltaico: una capacità di produzione diffusa e principalmente prodotta da fonti rinnovabili. Piccoli impianti eolici, impianti mini-idroelettrici, caldaie di cogenerazione: queste sono le prospettive che l'industria innovativa, quella che respinge i monopoli e si rimbocca le maniche, ci propone. Ma perché questo avvenga serve ammodernare la rete, passare dal modello fordista di distribuzione dell'energia, fondato sulle grandi centrali, ad un modello a rete, diffuso, capace di compensare i picchi. Il consumo elettrico segue l'organizzazione della società: di fronte al ridimensionamento degli impianti produttivi e ad una società che sempre di più si fonda sui servizi, il concetto di piccolo diventa anche efficiente. Terziario e consumi domestici, cioè le tipologie di consumi che si possono orientare allo scambio sul posto, corrispondono a circa la metà del consumo energetico nazionale. Le centrali che già ci sono basterebbero ampiamente per coprire i consumi dell'industria. Per costruire una centrale a gas servono tre anni di lavoro e le tecnologie e le imprese che lavorano sui componenti ad alto valore aggiunto sono in larga parte straniere. Per installare un piccolo impianto a fonte rinnovabile servono poche settimane e le tecnologie o sono tedesche o sono italiane. Se solo il conto energia sul fotovoltaico avesse goduto delle risorse destinate nel 2005 alle fonti assimilate, avremmo avuto tanta energia quanta ne consumano Abruzzo e Calabria messe insieme. Questa è, sul mercato elettrico, la vera liberalizzazione: rendere tutti potenziali produttori attraverso fonti ad impatto zero. Già nel provvedimento che oggi voteremo ci sono le premesse di questo modello: promuovere le associazioni di consumo, dando piena attuazione alla direttiva europea, significa costruire quello zoccolo su cui poggia una produzione diffusa. Certo, questo non basta: serviranno interventi e investimenti, soprattutto sulla rete. Ma il cammino comincia ora. Oggi approveremo un provvedimento di estrema importanza, atteso dalle famiglie e positivo per l'ambiente, dove i criteri di necessità e urgenza sono assolutamente evidenti. Ed è per tutto questo che, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani,

Signor Presidente, colleghi senatori, già ci siamo confrontati sui presupposti di costituzionalità di questo provvedimento. Oggi vi è la necessità di un voto unanime sul punto di merito. La direttiva del Parlamento europeo, recepita da questo atto Senato, fissava un termine preciso, quanto breve, per la liberalizzazione del mercato energetico anche ai clienti domestici. Ora, mancando nella legislazione italiana una specifica regolamentazione per tale passaggio, è imprescindibile colmare questa lacuna, dettando una normativa certa e definita a tutela degli utenti domestici. In tal modo - nell'ottica del completamento del processo di liberalizzazione avviato - la disciplina in esame, punta su due obiettivi corretti e mirati: contenere misure di avvio del mercato per i clienti finali in tema di erogazione di energie elettrica e gas naturali; mantenere sempre misure di garanzia a tutela delle famiglie in modo che la scelta tra nuove offerte e mantenimento del fornitore attuale possa avvenire senza il rischio di subire aumenti. Tuttavia, la bontà (ovvero l'interesse positivo) di questo provvedimento è legato anche ad altre regole generali, laddove sanciscono regole funzionalmente connesse alla completa apertura del mercato, quali la separazione funzionale e gestionale dei sistemi elettrico e gas naturale dalle altre attività non direttamente connesse; l'effettiva indipendenza e trasparenza gestionale, l'incremento di politiche concorrenziali specialmente nelle forniture, la separazione tra attività di vendita e di distribuzione all'utenza, mantenendo *standard* stabiliti di rapidità e di adattamento. In particolare e - nel concludere - ribadisco l'importanza di dare attuazione alle disposizioni oggetto di voto, che volge uno sguardo attento alle famiglie con l'intento di consentire una scelta libera, non condizionata da eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi. Per questo motivo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sinistra democratica voterà a favore di questo provvedimento le motivazioni in questa mia breve dichiarazione di voto, avendo già avuto modo di intervenire più diffusamente nel corso del dibattito generale, dove ho avuto modo di esplicitare i punti di consenso sul decreto

che è servito a migliorare ulteriormente i contenuti di questo decreto, con l'apporto di tute le forze politiche. Mi rendo perfettamente conto che sarebbe stato meglio se in quest'Aula avessimo potuto affrontare i contenuti di questo decreto-legge nell'ambito di una discussione più generale, affrontando appunto la legge delega sull'energia e il gas naturale, il disegno di legge n. 691, che già da qualche tempo è in attesa di essere discusso e mi auguro che ciò avvenga in tempi più rapidi possibili. Ho sentito che probabilmente lo faremo a settembre. Mi auguro che questa volta il calendario venga rispettato. Ritengo però che oggi risulti chiaro a tutti che è necessario approvare questo decreto-legge per introdurre quelle misure volte a tutelare il consumatore finale, ad impedire l'aumento ingiustificato delle tariffe e a mantenere inalterati i livelli di tutela previsti nelle norme comunitarie, che definiscono il trattamento dei clienti finali rimasti di fatto nel mercato vincolato. Ciò avviene perché, come è già stato detto, la legge n. 239 del 2004 introduce la scadenza del 1° luglio, senza stabilire regole e regimi di tutela per i clienti finali. Di conseguenza, per evitare sanzioni da parte della Comunità Europea e contenziosi da parte degli utenti, il Governo si è giustamente deciso a proporre questo decreto-legge, le cui norme si prefiggono lo scopo di sviluppare la concorrenza, di tutelare il consumatore nella fase di transizione fra il vecchio e il nuovo regime e rendere consapevole ed informata la scelta da parte dei consumatori da diversi punti di vista, non ultimo certamente dal punto di vista dell'impatto ambientale. Lo sviluppo della piena concorrenza è favorito dagli intenti in merito alla separazione delle reti dalla gestione del servizio e alla non discriminazione all'accesso delle informazioni da parte delle società di distribuzione verso le società di vendita.

le strade da intraprendere per ottenere tale difesa, in modo che il consumatore non venga danneggiato da ingiustificate modificazioni delle condizioni contrattuali e da aumenti dei prezzi. Il lungo *iter* del disegno di legge delega n. 691 in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia e del gas naturale non ci ha portati a definire in tempi utili il provvedimento. Ciò ha prodotto una situazione di infrazione con la Comunità europea che rischia di trasformarsi in sanzione: non convertire oggi il decreto-legge produrrebbe gravi danni per i cittadini, in questa fase di passaggio da un mercato vincolato ad un mercato libero. Per queste ragioni e per quelle esposte durante il mio intervento nel dibattito generale la Sinistra Democratica voterà a favore di questo provvedimento per convertire il decreto in legge e dare così piena attuazione ai suoi contenuti,

Signor Presidente, colleghi, anche se questo provvedimento va incontro ad una richiesta di adeguamento alla normativa europea

spende annualmente di energia 700-800 euro in più di una famiglia francese, se è vero che i costi per l'industria dell'energia sono sempre di gran lunga superiori ai *competitor*, alle industrie che competono e che sono grandi consumatrici di energia sul mercato europeo, noi speriamo veramente che qualcosa avvenga. Dal 1° luglio si esce dal vecchio sistema delle tariffe e si passa a bollette calcolate sommando prezzi e tariffe. Il prezzo dell'energia, pertanto, sarà determinato liberamente dal mercato tramite le offerte delle diverse società di vendita. Restano invece soggetti a tariffe delle autorità le altre voci e cioè i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, che necessitano peraltro di infrastrutture e non possono essere messi in concorrenza, e gli organi generali di sistema già citati. La nuova bolletta, dunque, sarà composta, oltre che dalle imposte, da un prezzo dell'energia e da una tariffa per i servizi legati alle infrastrutture e alle connessioni. Nel mercato libero le imprese di vendita al dettaglio acquistano l'energia elettrica all'ingrosso per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per il pagamento del servizio e garantiscono ai clienti le prestazioni commerciali indicate nel contratto. Il distributore, da parte sua, continua ad assicurare che il trasporto dell'energia sulla rete avvenga con continuità ed efficienza, fino al contatore incluso, e interviene in caso di guasto agli impianti per portare l'energia alle case. Il 2006, peraltro, sarà ricordato come l'anno più caro per i prodotti energetici. Infatti, sia a causa dell'aumento del petrolio sia per le carenze strutturali dei il nostro Paese è purtroppo uno dei peggiori, sia per la mancanza di un serio piano energetico basato sui risparmi e le fonti alternative sia inoltre per la mancanza della razionalizzazione del settore della distribuzione e della vendita dei carburanti nei centri commerciali, si è determinato per ogni famiglia italiana un aumento spropositato.

con serietà il discorso del costo energetico per il Paese, dobbiamo farlo a tutto campo, smettendola di raccontare bugie sulle energie alternative ma senza per questo

uno sguardo sincero e convinto per il futuro di questo Paese.

per la grande occasione mancata, con questo disegno di legge insufficiente e poco coraggioso, di tentare di risalire la china che in Europa ci vede sicuramente tra gli ultimi anche in questo settore. un'occasione formidabile, anche perché l'Unione europea da molti anni ha indicato la strada e, soprattutto, un piano energetico molto preciso e abbastanza cogente, aiutandoci a compiere delle scelte mirate, non nuove né solitarie, ma coerenti con quanto stanno facendo, o hanno già fatto in molti casi, i Paesi europei. Grande delusione, dicevo, soprattutto per l'aver mancato l'obiettivo principale che l'Unione si pone, cioè quello di creare un mercato unico europeo dell'energia basato su alcuni punti cardine sui quali, purtroppo, questo disegno di legge è profondamente latitante: innanzi tutto il coraggio di alcune scelte che il mutare dei tempi e anche l'evolversi delle tecnologie dovrebbero indicare ai legislatori, prima tra tutti la legge che impone di sapersi anche pentire di scelte sbagliate e di saper adottare i correttivi necessari. Alludo alla raccomandazione contenuta nel piano dell'energia europea per quanto riguarda il limite da porre alla dipendenza dalle importazioni e soprattutto dal petrolio e quindi il coraggio di ammettere che il bando a suo tempo emesso nei confronti dell'utilizzo del carbon fossile fu forse un momento errato di caccia alle streghe. Oggi nuove tecnologie e nuove capacità di reperimento di questa materia prima consentono di guardare di nuovo al carbon fossile come ad uno dei famosi mali minori al confronto con i danni ambientali che sicuramente l'uso del petrolio e degli oli provoca. C'è anche una mancata presa di coscienza di una revisione coraggiosa, che altri colleghi hanno ricordato, del bando che anche nel nostro Paese, in particolare nel nostro Paese, fu posto nei confronti dell'energia nucleare. Si è celebrata quest'anno la festa per i primi 50 anni del Trattato Euratom, vi è stato al Parlamento europeo un momento solenne di riconsiderazione ma anche di rilancio di questa proposta, che non è soltanto tecnologica: ebbene nessuno ha ribadito o ha rilanciato la caccia alle streghe, la volontà di chiudere questa esperienza ma, viceversa, se ne é sottolineata la validità soprattutto per quanto riguarda il minore impatto ambientale rispetto ad altre materie prime. Naturalmente, anche in questo caso, la garanzia della sicurezza è prioritaria e la tecnologia che è cambiata e si è evoluta può aiutare a compiere scelte nuove e coraggiose, tanto più che tutti sanno che con il nucleare noi dobbiamo convivere in quanto è una libera scelta che ciascuno Stato europeo può adottare: come noi abbiamo detto no altri continuano ad impegnarsi con il loro voto favorevole e, in questo momento, in Europa vi sono più di 150 reattori: non a caso l'energia nucleare copre il 36 per cento del nostro fabbisogno. C'è ancora una grande delusione, in questa legge, per quanto riguarda il raggiungimento, o quantomeno l'avvicinamento, dei due grandi obiettivi, direi quasi ideali, che ci si sta prefiggendo: quello di raggiungere, entro il 2020, una riduzione dei consumi cento, almeno per quanto riguarda il petrolio, e del 30 per cento per quanto concerne la produzione di gas serra. Sono impegni che altri Paesi stanno già assolvendo e stanno già raggiungendo. Noi siamo molto lontani. Dei dieci punti previsti dal piano europeo per l'energia noi forse, in questo momento, saremmo in grado di assolverne un paio al massimo. Quindi, la liberalizzazione del 1° luglio non dico sul nulla, ma su ben poco: è fatta, come si usa dire, soprattutto sulla carta piuttosto che su concrete basi giuridiche tecniche e soprattutto politiche. La distanza tra produttori, distributori e clienti finali, sia domestici che non, nel nostro Paese è ancora abissale. Così come ha ragione chi ha gridato poco fa, mi pare il collega Stefani, che anche il richiamo alle energie alternative, alle energie rinnovabili, è bello, è romantico ma è ancora una volta un'utopia che noi non ci possiamo ancora permettere, a differenza di altri paesi che ne hanno già fatto, viceversa, una fase credibile del loro approvvigionamento energetico. Noi abbiamo anche qui un obiettivo da raggiungere, quello del 20 di energia rinnovabile entro il 2020. Bene, molti Paesi hanno già raggiunto questo traguardo, noi oggi siamo circa al 7-8 per cento, colpa anche di una mancanza di convinzione nel finanziare seriamente la ricerca scientifica e tecnologica; 150 milioni di euro all'anno sembrano tanti, ma, in realtà, se vogliamo realizzare questi obiettivi ambiziosi, non sono tanti, sono pochissimi. Siamo ancora indietro anche nella ricerca per quanto riguarda le tecnologie, i ritmi e, soprattutto, la convinzione nel battere strade nuove. Come per noi è utopia raggiungere quel 20 per rinnovabili nel 2020, è davvero utopia immaginare di scrollarci di dosso la dipendenza dai fornitori che vengono da lontano; la Norvegia, l'Algeria, la Russia, per quanto riguarda il gas. Il richiamo alla solidarietà tra Stati dell'Unione Europea ha anche questo scopo e in caso di crisi, che abbiamo vissuto anche in epoca recente, la solidarietà ci aiuterebbe a limitare i danni e i disagi in caso - diciamolo tra virgolette, ma è una realtà - di «capricci» del fornitore o di forzature; quando anche noi rischiammo, lo ricorderete, di rimanere a secco di gas per certi rubinetti che non venivano più aperti. Questa solidarietà darebbe maggior morale oltre che maggior possibilità di sopravvivere anche all'Europa. Quindi, solare, eolica, energia fotovoltaica, utilizzo delle biomasse, sono belle immagini che ci diamo, di cui ci circondiamo, ma sono ancora esperienze che vengono limitate, che appartengono a poche Regioni particolarmente progredite. Eppure, è in queste immagini che sbagliamo per impegnare la nostra fantasia e per concentrare anche iniziative legislative come questa, mentre dovremmo affrontare più seriamente altre risorse, altri nodi e, soprattutto, avere più coraggio nel dire alla gente che una gran parte delle possibilità di fronteggiare le difficoltà energetiche deriva dalla capacità di di consumare di meno, quindi, di risparmiare. Anche questo, signor Presidente, nel disegno di legge che stiamo discutendo è detto in maniera assolutamente insufficiente. Per tale ragione confermo il voto contrario del mio Gruppo

intervengo brevemente per sottolineare ancora una volta l'incoerenza di questo Governo che a parole si professa favorevole alle liberalizzazioni e poi nei fatti adotta provvedimenti che contraddicono in gran parte la finalità per cui sono adottati. Questo decreto‑legge rappresenta un ulteriore esproprio nei confronti del Parlamento su un tema così importante quale l'energia. La Commissione Attività produttive ha lavorato con serietà e impegno fin dalla presentazione del disegno di legge n. 691 e ha apportato notevoli miglioramenti al testo presentato dal Governo, frutto di un discussione anche accesa, ma corretta tra le varie posizioni, presentando alla fine in Aula un testo che esprimeva la volontà del Parlamento sul tema. Questa volontà è stata più volte tradita, già con la scorsa finanziaria che ha scorporato parte delle misure contenute nel disegno di legge, e viene tradita anche oggi con questo decreto-legge che sottrae al testo un'altra parte importante del suo contenuto.

Questo disegno avrebbe invece permesso di affrontare e risolvere le questioni in oggetto con gli strumenti adeguati e nei tempi previsti. Sappiamo bene che sono ancora una volta le contraddizioni e le posizioni inconciliabili all'interno della maggioranza che hanno impedito l'approvazione del provvedimento. Contestiamo quindi in radice la scelta di adottare un decreto-legge, che diminuisce ulteriormente il margine decisionale del Parlamento su temi così importanti e su cui non si può procedere con queste modalità. Ma anche dal punto di vista del contenuto vi sono misure per cui non sussiste il requisito della necessità e dell'urgenza quali quelle in materia di stoccaggio del gas, che non si capisce bene quale attinenza abbia con la scadenza relativa all'apertura del mercato elettrico per gli utenti finali, prevista dalle norme europee. Abbiamo inoltre qualche perplessità su come questa liberalizzazione viene attuata: perché se apertura del mercato vuol dire concorrenza non ravvisiamo la necessità e la coerenza della misura che attribuisce all'Autorità per l'energia, come bene ha detto il collega della Lega, di fissare prezzi di riferimento, misura che ci sembra in contrasto con una vera liberalizzazione che per sua natura esige una libertà nella fissazione dei prezzi. Piuttosto, una tutela effettiva dei cittadini poteva essere assicurata da obblighi informativi diretti a rendere confrontabili le varie offerte presenti sul mercato. Temiamo che anche queste liberalizzazioni siano solo di facciata ma poco di contenuto. Come del resto abbiamo sottolineato in occasione degli altri interventi di questo Governo sulle liberalizzazioni, è evidente che i condizionamenti esistenti all'interno della maggioranza impediscono di adottare misure che vadano effettivamente nella direzione di liberalizzare i mercati. Brevemente vorrei anche mettere in evidenza che, come accaduto in molte altre occasioni, il lavoro della Commissione è stato del tutto disconosciuto. In Commissione, infatti, all'unanimità era stato approvato un emendamento, presentato da me e dal collega Ruggeri a nome del mio Gruppo dell'UDC, che migliorava il testo e rendeva il mercato dell'energia elettrica realmente liberalizzato rendendo non obbligatori i prezzi di riferimento determinati dall'Autorità, ma questi dovevano essere semplici punti di riferimento a fini informativi per i clienti-consumatori. Altro che liberalizzazioni, qui abbiamo qualcosa che assomiglia a delle vere e proprie tariffe amministrate. La contraddizione è evidente: come si possono conciliare prezzi di riferimento obbligatori e liberalizzazione del mercato? Vorrei proprio che il Governo ce lo spiegasse. Evidentemente ci sono state pressioni per cambiare la disposizione di assoluto buon senso, e - ripeto - adottata all'unanimità dalla Commissione. Questo fatto, che di per sé è molto grave perché vanifica il lavoro della Commissione, dimostra la debolezza di questo Governo che cambia idea a distanza di breve tempo e soprattutto dimostra la mancanza di chiarezza e unità nella sua linea politica, sia che si tratti, come in questo caso, di energia, sia, più in generale, come è successo la scorsa settimana, di politica economica. Per queste ragioni, nonostante la condivisione di alcuni punti e soprattutto della finalità del provvedimento, che però viene per molti aspetti negata nei contenuti, esprimo, a nome dell'UDC, la nostra contrarietà all'approvazione di questo decreto-legge.

credo che non sfugga a nessuno la centralità della questione energetica, che è oggettivamente la questione del nostro tempo. Essa si intreccia al centro di tutte le crisi internazionali, si intreccia con la prospettiva di un decadimento ambientale, con la grande questione del clima. Tutte questioni e problemi che non possono essere assolutamente affrontati e risolti in termini nazionali. Da qui credo che venga la convinzione che noi dobbiamo riuscire, con l'Europa, ad avere una voce comune per risolvere le questioni dell'energia sotto i profili

Questi sono i nodi che abbiamo di fronte. Il primo impegno è quindi di fare dei passi insieme, in comune, con l'Europa e questo decreto si pone, come primo obiettivo, quello di rispondere e di risolvere la questione sollevata da un'infrazione a livello europeo. Certamente è un tratto, solamente un tratto della questione di come si può affrontare nel complesso la questione energetica, ma è un primo passo importante e si muove innanzi tutto sul terreno delle liberalizzazioni, che ci viene dettato dall'Europa, ma che può essere efficace solamente se viene vista, soprattutto in questa fase, come superamento della logica dei campioni nazionali, in un'ottica però che eviti la ricostituzione di posizioni dominanti e quindi non come consegna delle grandi scelte definitivamente e completamente al mercato, ma in termini di superamento dei vincoli che impediscono in Europa di assumere una posizione forte su questo terreno. Nel momento in cui si apre alle liberalizzazioni, si pone immediatamente il problema di far sì che questo processo salvaguardi non solo gli utenti, ma anche i territori deboli e quindi di inserire i giusti contrappesi che possono consentire di proseguire su questo percorso senza provocare problemi di natura sociale. Su tale problematica abbiamo avuto un confronto serio in Commissione. Ho ascoltato l'intervento del senatore Maninetti e anch'io ritengo che abbiamo svolto un buon lavoro in quella sede; mi sembra però che le posizioni che lì sono emerse, indipendentemente dal testo letterale che poi è passato, diano contezza del ragionamento e del confronto che abbiamo avuto proprio sulla qualità specifica e sulle modalità con cui andavamo ad approvare il processo di liberalizzazione. Abbiamo previsto l'obbligo di inserire nell'offerta un prezzo di riferimento, ma nessuno può impedire ad una società di presentare offerte migliorative. Quindi, l'effetto del mercato mercato nel confronto tra le varie offerte può essere mantenuto, perché il prezzo di riferimento può e deve essere inteso esclusivamente come un tetto da non superare; quindi, non cancella la possibilità della concorrenza tra le varie offerte.

stata prodotta una determinata energia è una spinta ad un consumo critico avanzato, che può essere un altro motore per l'avanzamento verso gli obiettivi che ci vengono dettati in sede europea. Non si tratta solo di questioni etiche: credo sia importante, di un sistema di solidarietà orizzontale tra i vari territori e anche verticale nei confronti delle generazioni, affrontare il problema dell'aumento delle temperature. Oggi la questione delle fonti energetiche alternative e rinnovabili è anche una grande opportunità economica, perché i ritmi di sviluppo dell'economia di India e Cina non consentono assolutamente di continuare ad osservare

riuscire a far sì che l'Europa parli su questo terreno con una voce sola. Certo, dobbiamo avere il senso della misura: il decreto in conversione e stato dettato dall'urgenza e dal bisogno immediato di rispondere ai temi sollevati dall'inflazione, e lo abbiamo fatto;

fa dal senatore Allocca. In Commissione si è lavorato bene, si è lavorato in modo aperto, senza pensare ai rispettivi schieramenti, soffermandosi sull'esame dell'evidenza dei fatti e delle questioni che esaminavamo. esaminavamo. C'è stato un lavoro intelligente e c'è stata disponibilità, da parte del relatore, ad accogliere tesi inizialmente diverse.

avessero continuato ad agire con la stessa coerenza e la stessa disponibilità. Ma quando abbiamo assistito, nonostante l'interruzione, alla - perdonatemi i termini - protervia e all'arroganza di voler far rispettare qualche *diktat* esterno a questo ramo del Parlamento, la situazione è cambiata. Non ci siamo, non ci siamo assolutamente.

per i richiami ricevuti dalla loro Capogruppo. Immagino che il senatore Barbieri, simpaticissimo collega campano, non abbia ricevuto analogo rimprovero per l'emendamento precedente

però che senatori, colleghi, persone serie che in Commissione hanno votato in un certo modo debbano poi subire in Aula il *diktat* che non si possono accettare cambi,

sistema di problemi, di articolazioni, di strutture. Possiamo facilmente scivolare dalla considerazione di questo particolare provvedimento alle alle tematiche più generali. Cercherò di evitare questo facile diversivo per concentrarmi invece sul tema alla nostra attenzione.

le sue disposizioni sono addirittura tipiche di un regolamento più che di una direttiva inevitabilmente a maglia larga, come dovrebbero essere le direttive europee che si rivolgono In molti casi, ed in particolare in questa direttiva, alcune disposizioni sono a maglia molto stretta e addirittura presentano caratteristiche di un'attività regolatoria.

e poi ci siamo dimenticati delle prescrizioni di cui all'articolo 15, che prevedevano l'impegno del Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per far sì che le minuziose disposizioni della direttiva comunitaria in questione

Esse infatti vengono incontro alla necessità del superamento di una procedura d'infrazione molto ben precisata con cinque particolari rilievi

la maggior parte delle disposizioni in esso contenute rispetta i principi di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dalla Costituzione. per ricordare che si tratta di provvedimenti validi di tutela del nostro ordinamento nel campo energetico. Al comma 1 si stabilisce che le imprese di vendita dell'energia elettrica devono essere separate da quelle di distribuzione. Trovo corretta questa disposizione, perché è giusto che i monopoli naturali, come sono le imprese di distribuzione, siano trasparenti, non vincolati, né legati ad esigenze di mercato, liberi quindi per tutti coloro che utilizzano una infrastruttura fondamentale. In questo modo,

Ugualmente, condividiamo le prescrizioni di cui all'articolo 2, che tutelano i clienti domestici nel difficile passaggio della piena liberalizzazione del mercato, consentendo, ad esempio, la recessione dal

di fissare condizioni *standard* di erogazione del servizio. Non sono e non siamo assolutamente d'accordo sul mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di fissare, almeno transitoriamente, prezzi di riferimento per l'energia elettrica, sia perché si tratta di una disposizione che in questo caso non mi pare così allineata con il requisito costituzionale della straordinaria necessità ed urgenza, sia perché in effetti

essere tutelati se non hanno fatto la loro scelta del fornitore di energia elettrica. Siamo altresì d'accordo sulle disposizioni di cui al comma 5, che prevedono l'inserimento nella fattura delle imprese di vendita dell'energia elettrica di alcuni dati importanti quali l'indicazione delle fonti energetiche nel *mix* della fornitura di energia

all'attuazione di un precedente decreto del Ministro delle attività produttive del marzo 2006, che consente l'utilizzazione di imponenti risorse per la ricerca e lo sviluppo

tra l'altro, ad uno dei principali centri di ricerca italiani, il CESI Ricerche SpA, di procedere con la sua attività di ricerca sul sistema elettrico, bloccata dall'inizio del 2006.

ad una certa diffidenza espressa nei confronti del mercato elettrico e all'adozione di alcune - poche, per fortuna - disposizioni non pienamente allineate con i requisiti necessari per l'inserimento in un decreto-legge. Penso, ad esempio, alla disposizione 1, che prevede la separazione funzionale dell'unica impresa che lavora nel campo dello stoccaggio del gas, la Stogit spa.

che ha dato un grande contributo alla creazione di un clima positivo all'interno della Commissione stessa. Esprimo altresì apprezzamento per l'azione emendativa intrapresa sia in Commissione, sia in

nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo su questo provvedimento, sottolineo in modo particolare il fatto che che non si tratta di un provvedimento al di fuori di un disegno complessivo, ma, anzi, si tratta di un ulteriore tassello alla politica che il Governo sta perseguendo con molta determinazione dall'inizio della legislatura, con tre obiettivi ben definiti. Il primo obiettivo è quello di togliere ingessature e incrostazioni al sistema Italia. Ve ne sono molte e sono molto resistenti; il sistema Italia ha invece bisogno di essere alleggerito. Il secondo obiettivo è offrire nuove opportunità, in modo particolare per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro,

dei mercati protetti (particolarmente nel settore dei servizi), che sono un ulteriore peso che il sistema produttivo italiano deve sopportare. Con questo provvedimento si completa l'azione nel settore dell'energia elettrica, arrivando alla piena attuazione di una liberalizzazione in tutta la filiera, dalla generazione al mercato all'ingrosso, al mercato al dettaglio, fino a tutti i clienti finali. Devo ricordare, tra l'altro, che in questo settore, a differenza di quanto è avvenuto per il gas, è già stata trovata una soluzione adeguata per assicurare l'indipendenza della rete e, quindi, uno dei meccanismi fondamentali per la realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale.

con i primi provvedimenti Bersani-Letta, e che è proseguito nella scorsa legislatura, mi permetto di dire, a nostro avviso, con qualche eccesso di timidezza (però il cammino era proseguito); tale percorso giunge ora a compimento con questo decreto-legge. Possiamo dire che si è trattato solo di aspetti formali? Direi di no. Già si vedono e sono misurabili dei risultati importanti. Posso ricordare, ad esempio, che ad esempio, che ancora nel 2003, nel campo della generazione elettrica, il produttore principale copriva il 49,4 per cento della generazione; oggi questa quota è discesa al 34,8 Posso ricordare che nel 2003 i quattro maggiori produttori coprivano i due terzi dell'intera produzione; oggi questa percentuale è scesa a poco più del 65 una concorrenza più elevata, che comincia ad avere effetti anche nel campo dei prezzi. Certo, l'energia in Italia, per molti motivi, ha dei costi elevati, più elevati della media europea, particolarmente nel campo dell'energia al servizio del settore produttivo,

È stata presentata un'indagine della Camera di commercio di Milano che dimostra come nell'anno precedente i clienti liberi, rispetto a quelli vincolati, sono riusciti a spuntare risparmi che si aggirano tra il 16 e il 9 per cento, a seconda della classe di consumo dell'energia elettrica. Si tratta quindi di risultati che cominciano ad agire anche nel portafoglio dei clienti domestici ed industriali. Naturalmente, creare le condizioni giuridiche per una piena concorrenza non significa averla già raggiunta. Con questo provvedimento completiamo il quadro delle norme che consentono di realizzare un mercato aperto, ma molto deve essere fatto perché diventi realtà. Basti pensare che già prima della scadenza del 1° luglio esisteva in Italia un mercato aperto: erano circa 7,6 milioni i clienti che erano diventati idonei con la precedente riforma, cioè potenzialmente liberi di cercarsi un proprio fornitore. Ma solo il 9 per cento di questi ha utilizzato la possibilità di andare a trovare, sul piano del prezzo e della qualità del servizio, il fornitore ritenuto migliore. Come è stato ricordato, il decreto necessariamente individua un regime transitorio per accompagnare sul mercato un processo molto complesso che riguarda categorie di forniture agevolate per motivi sociali o perché riguardano piccoli produttori che potrebbero ricavare un danno da un'apertura improvvisa del mercato e che devono essere accompagnati per poter usufruire fino in fondo dei vantaggi, in termini di prezzo, che l'apertura del mercato potrà portare con sé. Occorre poi ulteriormente lavorare per una diversificazione dell'offerta, in modo che in tutte le aree del Paese vi sia un mercato concorrenziale, perché attualmente questo ancora non si è pienamente realizzato. realizzato. Occorre ancora lavorare per investire sulla rete, sulla sicurezza generale del sistema, su una più forte integrazione a livello europeo. Non c'è dubbio che un mercato ben funzionante porterà vantaggi crescenti per i consumatori; tuttavia, non possiamo trascurare un fatto che riguarda la precarietà, la delicatezza del nostro sistema energetico. Noi abbiamo un bilancio energetico complicato. Sappiamo che solo il 15 per cento del nostro fabbisogno energetico è soddisfatto da fonti nazionali: in parte l'autoproduzione, peraltro calante, del gas e di un po' di petrolio, e in parte fonti rinnovabili, però in gran parte concentrate nell'idroelettrico, quindi figlie del grande ciclo di investimenti realizzati tra la fine dell'Ottocento e il Novecento. Tutto il resto - gas, carbone e

per il gas e il petrolio, con problemi di acquisto in aree geopolitiche spesso non del tutto stabili.

potuto sviluppare anche le politiche che si sono impostate per mettere in maggiore sicurezza il sistema energetico - aver puntato sul gas e significa lavorare perché il sistema sia più sicuro: quindi, diversificazione delle fonti, potenziamento dei dei gasdotti, possibilità di realizzare rigassificatori che rendono maggiormente indipendente il sistema. Possiamo dire, comunque, che si raggiunge un risultato importante. Termino con una riflessione che riguarda il lavoro del Parlamento. Anch'io devo riconoscere che è stato fatto un lavoro importante in Commissione e ringrazio il relatore, il Presidente e l'opposizione per il contributo che hanno dato ai lavori. Questo Questo decreto si è però reso necessario perché il provvedimento presentato dal Governo il 28 giugno del 2006 alla data odierna ancora non è stato approvato da un ramo del Parlamento. Ciò pone un grande problema di funzionalità della sede parlamentare su cui tutti - maggioranza e opposizione - dobbiamo lavorare, perché alla fine la credibilità dell'istituzione parlamentare sta in capo alla capacità di dare soluzione rapida ai problemi del Paese. Buone leggi, ma tempestive! Credo che questo sia il segnale che dobbiamo ricavare anche dal lavoro positivo fatto in Commissione

*(Aut)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Per le Autonomie, annuncio il voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73. In effetti, la mancanza di regole e di regimi di tutela dei clienti finali del mercato dell'energia elettrica non poteva che sollecitare il Governo all'emanazione di un decreto-legge, atteso, da un lato, allo spirare del termine del 1° luglio 2007 per la liberalizzazione del mercato medesimo e verificato, dall'altro lato, il mancato compiersi dell'*iter* parlamentare nel disegno di legge n. 691, già approvato dalla competente nostra Commissione, ma non ancora approdato all'Aula. Abbiamo in proposito appena appreso la determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi di farne slittare la trattazione in Aula al prossimo settembre. C'erano dunque tutte le motivazioni per la decretazione d'urgenza, anche con riferimento alla puntuale attenzione della Commissione europea, al corretto trattamento da riservarsi ai clienti finali ed il rischio di avvio della procedura di infrazione. Per questo motivo, il Gruppo ha stamani ritenuto di non condividere taluni rilievi in merito, contenuti nell'intervento del collega Possa. Con questo decreto si introducono disposizioni urgenti di valenza, anche transitoria, e quindi integrabili e migliorabili, secondo criteri che il Parlamento volesse poi valorizzare in fase di approvazione del disegno di legge n. 691. L'obiettivo principale del decreto è quello di accettare la completa liberalizzazione del mercato in una prospettiva, però, di passaggio graduale. Credo possano giustamente esprimere soddisfazione le associazioni dei consumatori, nel senso di poter verificare nei primi mesi l'identità dei distributori, di poter confrontare le loro offerte, di poterle verificare rispetto alle tariffe di riferimento. Risulta importante, a questo proposito, il ruolo dell'Autorità indipendente, della quale potremmo anche noi chiedere l'integrazione nella composizione, avendo ascoltato l'intervento del senatore Polledri circa i minimi termini raggiunti proprio dalla composizione di quell'organismo. Per il cliente finale l'obiettivo è quello di poter sottoscrivere in piena scienza un contratto garantito da norme di trasparenza scegliendo il proprio distributore. Su questa linea di indirizzo si muove l'articolazione del decreto, anche nelle disposizioni di maggiore complessità. Penso al comma 1 o al comma 3. Credo che la Commissione abbia effettivamente compiuto un buon lavoro ma valuto anche positivamente gli emendamenti introdotti dall'Aula, che rendono in taluni punti più stringenti le iniziali previsioni. Non è discutibile l'opzione decisa del Governo verso la liberalizzazione del mercato, peraltro opportunamente temperata da elementi di garanzia per gli utenti, chiamati a misurarsi con una prospettiva di scelta in concorrenza, anche a livello domestico. Con questo decreto si conferma una strada precisa, con un completamento dello scenario generale del comparto energetico che dovrà essere integrato con passaggi legislativi e con l'adeguata operatività di controlli progressivi da parte della citata Autorità. Confermiamo il nostro voto favorevole.